dei beni e delle attività culturali e del turismo, onorevole Dario Franceschini, risponderà a quesiti sui seguenti argomenti: assetti organizzativi del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo nonché degli enti vigilati; iniziative per la promozione del turismo culturale. **Seguito della discussione del disegno

prima sull'ordine e poi sul disordine. Signora Presidente, voi avete dato lettura degli emendamenti e della relativa ammissibilità sugli emendamenti agli articoli del decreto‑legge; non credo - se non ho ascoltato male - di aver ancora sentito, invece, il parere rispetto agli emendamenti al disegno di legge di conversione, che non credo siano ancora stati enunciati. difficoltà - e credo che valga la pena di interessare anche il Presidente per la portata del problema

le ammissibilità e i contenuti di un decreto-legge sono stati fissati da una serie di sentenze della Corte costituzionale, al punto che sono stati costituzionalizzati nella riforma, che mi auguro comunque venga bocciata al *referendum*. abbiamo riscontrato l'ammissibilità di un emendamento sulla proroga di un termine rispetto alla decretazione legislativa (c'è qualche precedente, purtroppo anche dovuto a qualche nuovo nostro collega); ma quello che mi appare inverosimile è che venga accolto un emendamento, di natura assolutamente ordinamentale, che dà vita a una fondazione autonoma, denominata Fondazione dei Corpi della Croce rossa italiana; dopo di che si demanda la scrittura dello statuto, di cui si prevede quale sia l'aspetto ordinamentale, quali siano gli organi direttivi, quale sia il patrimonio e quale sia il personale, al punto che l'estraneità della materia è tale che vi è un «*Conseguentemente, al titolo del disegno di legge aggiungere, in fine, le seguenti parole: ". Costituzione della Fondazione dei Corpi della Croce Rossa Italiana"*». Non so cosa vi sia di necessario, urgente urgente e omogeneo rispetto al resto del contenuto. La prego veramente, signora Presidente, di fare un'approfondita valutazione e, nel caso, consultare anche il Presidente, perché se questi sono i principi

sul famoso emendamento 4.200, poi ritirato, ho cercato di informarmi rispetto al presentatore e ho scoperto che è il Governo stesso, che lo presenta e ne allega anche la relazione tecnica, da cui si evidenzia il contenuto di questo emendamento: è autorizzata per l'anno 2016 la cessione alla...

Credo, infatti, sia stata una sciocchezza averlo presentato e una sciocchezza averlo ritirato completamente. Posso capire nella parte in cui si assegnano quattro autovetture. Sulla marca e il modello ho qualche perplessità: due BMW 3018 a iniezione e due Volkswagen Passat 2.8;

lei vuole, facciamo passare i venti minuti sospendendo la seduta poi riprendo la parola su un altro emendamento; decida lei.

che il fatto di assegnare quattro automobili ad uso di intercettazione rispetto al terrorismo fosse una cosa necessaria, urgente e utile. Così come altrettanto inaccettabile è la lettera *b)*, che bene hanno fatto i relatori a ritirare, ma che vado a specificare perché nella relazione tecnica c'è anche quello: «in particolare 16 strumenti musicali per banda, di cui quattro filicorni, quattro tromboni, un sax, una tromba, un flauto e cinque clarinetti».

10.000 impermeabili per il Libano, 2.000 per l'Iraq, 12 fuoribordo, tre rimorchi, un'ambulanza, quattro gommoni, tre elicotteri, navi e motovedette, di tutto di più. Il significato è semplice:

Adesso, visti i risultati e i contenuti dell'emendamento, siamo andati per suonare e siamo stati trombati. Questa è la sintesi di quello che ho appena detto. Tuttavia, signora Presidente, la parte intervento rispetto al Governo è che se vuole rivedere - siamo ancora sul punto - la possibilità di attribuire quei mezzi, va benissimo, fatto salvo che poi bisogna stabilire in Somalia quali sono i terroristi e quali non lo sono. Prendiamola per buona e a lei invece assegno il compito, che mi sembra abbastanza scontato, di dichiarare inammissibile quell'emendamento.

della NATO, lo ritengo un atto pericoloso e inutile, non uso altri termini. L'unica cosa che mi meraviglia è che sia stato presentato dal senatore Sangalli, di cui ho un'enorme stima personale e politica, ma sono certo che non è farina del suo sacco. del suo sacco. È un problema serio, non capiamo a cosa stiamo andando incontro. Rischiamo seriamente, per una sciocchezza di questo tipo,

la vicenda Regeni è tutta da scrivere e da vedere per quanto inquietante e pericolosa, ma non c'entra assolutamente nulla. Tuttavia, vorrei dire che prendo atto che è avvenuto un fatto importante

Se si fosse rimesso all'Assemblea per la riforma costituzionale, per la legge elettorale e per tanti altri provvedimenti, ci saremmo certamente trovati a vivere cose migliori di quelle che viviamo. Naturalmente dico questo sapendo benissimo che il Governo ha voluto questo tipo di emendamento, anche se lo fa passare per una volontà

altrimenti cadiamo nel ridicolo e rischiamo cose serie. Sono allibito dal vedere come si gioca su argomenti così delicati per nulla. Ciò la dice lunga sull'improvvisazione e sul modo di essere

una barzelletta. Non ci stiamo rendendo conto di quello che è avvenuto e della serietà di un argomento come questo. Problemi di politica estera così delicati avrebbero meritato, con tutto il rispetto per i Sottosegretari, la presenza perlomeno del Ministro della difesa e del Ministro degli esteri.

Questo è il dato reale. Per cui, rimettiamo alla valutazione dell'Assemblea in tutta serenità e libertà la possibilità di riportare il testo alla prima stesura presentata dal Governo. Per tutto il resto ne parleremo nella dichiarazione di voto complessiva sul disegno di legge.

Sarà strumentale, però noi vorremmo capire l'ambito in cui ci stiamo muovendo. Capisco il dolore dei familiari, ma capisco meno quando si presentano al Parlamento europeo e chiedono il richiamo degli ambasciatori degli Stati membri dall'Egitto, la dichiarazione dell'Egitto come Paese non sicuro, la sospensione degli accordi di riammissione, degli accordi interforza, la sospensione degli accordi di fornitura di armi, degli accordi economici e il ritiro degli ambasciatori. Davanti a queste posizioni comprensibili per il dolore provato, ci troviamo adesso a discutere di un emendamento che non sposa queste tesi estreme, anche se nella sostanza è perché noi stiamo applicando una sanzione all'Egitto. Noi prendiamo uno di questi punti e in termini politici, diplomatici e culturali applichiamo una sanzione all'Egitto. tipo: cari egiziani, siccome secondo noi non collaborate, come dovreste, al caso Regeni, vi facciamo mancare i ricambi delle armi e degli aerei con i quali voi, nostri alleati, combattete il terrorismo. Questo è il messaggio che diamo. Abbiamo parlato di strumenti musicali, ma ci sono questioni forse più importanti di politica estera e il collega Gasparri ne ha fatto menzione. Noi siamo alle prese con problemi di questo tipo. Noi ieri abbiamo avuto il messaggio del Presidente del Senato, della Presidente della Camera e del Presidente dello Repubblica per rimuovere opacità per rimuovere opacità e situazioni di ombra di un fatto avvenuto trentasei anni fa che ci è costato 81 morti. C'è una vittima in Egitto; ci sono 81 vittime nel caso del DC-9.

felloni. Forse il Parlamento non lo sa, ma ne ho parlato come Ministro, come Governo italiano e nessuno mi ha smentito. Clinton ha scritto una lettera personale al presidente del Consiglio, Giuliano Chirac ha scritto una lettera personale in cui hanno chiamato fuori gli Stati Uniti e la Francia da quella vicenda. Hanno risposto 70 volte alle nostre rogatorie. Allora, scusate, se noi continuiamo, nell'immaginario collettivo, nella TV di Stato, a Bologna, negli sceneggiati, a dire che ci hanno ammazzato 81 persone,

che, dopo essere stati desecretati, però sono stati identificati con il simbolo di «segretissimo» e «segreto», quindi siamo a conoscenza di questioni di vitale importanza per andare a scrivere la verità su fatti di terrorismo che sono costati la vita a 81 persone,

nazionale? Con quale autorità ci rivolgiamo all'Egitto dicendo che applichiamo la sanzione e non forniamo più i pezzi di ricambio quando noi stessi, nei confronti degli italiani, dopo trentasei anni ci nascondiamo dietro il segreto? Ogni anno ci sono questi appelli solenni, ripetuti: ripetuti: contro ogni convenienza bisogna arrivare a scoprire la verità. Ma a chi la chiediamo la verità? Io lo so che è stata una bomba, lo sanno tutti, lo sa il Ministro degli esteri, il Ministro della difesa. Certo che non vanno a coprirsi di ridicolo con gli americani e i francesi con la storia della battaglia aerea. Ci sono le perizie mai

modo prendiamo in giro gli alti vertici dello Stato e loro prendono in giro gli italiani, se tutti gli anni di nuovo c'è questo rituale stanco sulla necessità vitale di arrivare a scoprire la verità su fatti così sanguinosi e gravi. Che risultato otteniamo invece con questa nostra improvvida iniziativa? Pensate che a livello internazionale passi inosservato - all'ISIS, ai gruppi terroristici, nel Medioriente - per quanto l'Egitto sta facendo (si veda quello che è successo ieri a Istanbul,

gli forniamo più i pezzi di ricambio, abbiamo già definito chi è l'assassino o chi copre l'assassinio: al-Sisi. Il Parlamento italiano ha già stabilito che loro sono i nostri nemici, sono quelli che hanno ammazzato un nostro cittadino. Credete che un emendamento di questo tipo non faccia il giro del mondo, che non sia un segnale di debolezza e di resa? A chi? *Cui prodest*? A chi può far piacere un emendamento di questo tipo che priva i nostri alleati della possibilità di intervenire anche a difendere noi? Il collega Gasparri giustamente l'ha ricordato: il terrorismo vuol mettere in ginocchio la Tunisia e l'Egitto dal punto di vista economico; i turisti non vanno più. È chiaro che rischia di diventare un'ulteriore polveriera perché anche l'Egitto può saltare per aria dopo la Libia.

o gli strumenti musicali - di ritirare questo emendamento per una questione di sicurezza nazionale, per una questione di coerenza. Per una volta facciamo un vero dibattito sui segreti, sulle stragi, su Ustica.

una marea di sentenze, e continua a ripetere del MIG libico che è caduto quindici giorni prima? Sono cose che non stanno né in cielo né in terra! Perché il Governo non viene a confrontarsi con il Parlamento? Perché non viene qui a dire quello che sa o quello che non sa? Perché non toglie il segreto o il segretissimo su quegli atti e ci permette di giudicare e di scoprire la verità? Noi non possiamo ribaltare sugli egiziani quelli che sono nostri difetti. Sono atteggiamenti - permettetemi - indecorosi sia per le istituzioni sia per gli italiani.

La durezza nei confronti dell'Egitto ci vorrebbe su altri piani. Ci sono accordi dell'ENI e accordi economici e, quindi, se volessimo dare delle risposte avremmo un campo infinito, ma vedo che alcune tematiche non vengono toccate.

In un momento di offensiva terroristica approvare un emendamento sui pezzi di ricambio degli aerei egiziani non ci sembra un atteggiamento particolarmente saggio e costruttivo,

non fa parte). Può darsi che su Cambridge e sui luoghi che hanno spinto Regeni a svolgere delle ricerche ne sappiano più di quello che hanno detto ai giornali. Stiamo però parlando di lotta al terrorismo. In tema di condanna di alcuni comportamenti possiamo calendarizzare mozioni dopodomani e discutere in Parlamento

per trasformare in ordine del giorno una proposta emendativa. In questo caso, non ho il potere di farlo, ma farei un invito analogo: studiamo uno strumento parlamentare che, senza arrecare danni ai rapporti bilaterali e alla sicurezza, lanci un monito. Questo sarebbe forse uno strumento più utile e confacente.

Signora Presidente, rinnovo anch'io il quesito posto dal collega Marton al Governo. È importante avere questo chiarimento, non soltanto per il Gruppo del Movimento 5 Stelle, ma per tutti quanti, in modo In questo caso specifico, il Movimento 5 Stelle dichiara il proprio voto favorevole all'emendamento 4.100/1, per motivi leggermente differenti rispetto a quelli che i colleghi in precedenza hanno evidenziato. Concordiamo in parte con il discorso fatto dal senatore Tarquinio:

che non rispettano i diritti umani. Non a caso su questo punto in Commissione c'è stata una discussione molto ampia. Noi abbiamo presentato il subemendamento 4.100/2,

Nel caso specifico, non possiamo fare a meno di dire che il caso Regeni per l'Italia ha rappresentato e rappresenta qualcosa di inaudito e di gravissimo. Siccome su questa vicenda ancora oggi non c'è

finalità dell'emendamento; non è detto che servano per combattere il terrorismo, perché questo non è specificato e noi non andremo a verificare se quegli aerei che si alzeranno in volo saranno utilizzati per combattere il terrorismo o per compiere altre azioni militari da parte dell'Egitto. Credo che sia

Palesemente, se si vota a favore di uno, bisogna votare contro l'altro, e viceversa. Noi voteremo contro l'emendamento 4.100/1 e a favore dell'emendamento 4.100 delle Commissioni riunite perché crediamo invece che sia giusto prendere atto della situazione che si è consumata nel corso di questi mesi. Vorrei ricordare ai colleghi non è che con questo emendamento rischiamo di creare una situazione di crisi con l'Egitto: noi siamo già in una situazione di crisi con l'Egitto, tanto è vero che ‑ lo ricordo a qualcuno che lo ha dimenticato ‑ abbiamo ritirato l'ambasciatore.

Vorrei però aggiungere un'altra riflessione, e lo dico anche al senatore Tarquinio con il quale spesso interloquisco positivamente, ma con il quale in questo caso, come si capisce, non sono d'accordo. Vorrei tentare di smentire un elemento di propaganda che viene raccontato,

questo supporto all'Egitto, non coglierebbe fino in fondo l'importanza della battaglia contro il terrorismo che quel Paese sta facendo.

F-16 in dotazione alle forze militari egiziane si dà il caso che nei mesi passati non siano stati utilizzati prevalentemente per attaccare le postazioni di Daesh le postazioni di Daesh ma, come peraltro il mio Gruppo parlamentare ha detto più volte presentando anche delle interrogazioni parlamentari in proposito, in particolare per attaccare Yemen e Siria attraverso operazioni militari unilaterali che l'Egitto ha fatto, non autorizzate dalle Nazioni Unite, che peraltro nei mesi scorso hanno ucciso anche alcune migliaia civili.

zona del mondo. Magari questi F-16 egiziani di cui stiamo parlando fossero impegnati semplicemente nella lotta contro Daesh. Qualche volta invece, anzi molto spesso, come si vede, vengono utilizzati per ipotesi di missioni non convenzionali, non coperte dall'ONU, peraltro anche con il frequente utilizzo delle cosiddette bombe a grappolo, messe al bando dalla Convenzione di Dublino. Quindi, mi pare che questo emendamento apra un mondo.

si fa «senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanzia pubblica», trattandosi di cessioni «già autorizzate da precedenti provvedimenti di proroga delle missioni internazionali». E conclude: «la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto, laddove erano previsti oneri per acquisto, ricondizionamento o trasporto nazionale ai luoghi di partenza, le relative spese sono state già sostenute

e al senatore Mario Mauro, per poi darla allo stimatissimo amico, il collega Caliendo, che ha comunque svolto un intervento. Signora Presidente, quest'Assemblea ha bisogno di equità.

abbiamo ricambi di magazzino. Capiamo perfettamente le motivazioni di chi dice che in questo momento storico è bene mantenere relazioni con la Repubblica Egiziana.

con le posizioni di politica estera dell'Europa e del nostro Paese. Premesso questo, a nostro avviso, armare o fornire

comporta indubbiamente dei rischi. Guardiamo non più come una foto statica, ma come un film, cosa è stato l'Egitto negli ultimi quattro anni,

colpo di Stato dei militari e oggi abbiamo un Governo presieduto da al-Sisi, che nei nostri confronti può dare relativa garanzia di stabilità. È finito? No. La fotografia è finita, ma il film continua. Ci possiamo fidare di uno Stato, di un Governo che ha avuto questo tipo di alternanze? E la nostra domanda rischiamo di armare e offrire dotazioni a Paesi che sono tutto fuorché stabili, *ergo* domani potrebbero essere utilizzate per scopi esattamente opposti a quelli che oggi pensiamo di ottenere? Con queste premesse, ribadiamo di avere tutto fuorché certezze: non ci sentiamo né di affossare questa tendenza ai rapporti

Comprendo il suo imbarazzo e, in qualche modo, la mia è una dichiarazione di solidarietà a suo riguardo. questo emendamento ha cercato di camuffare come una scelta, diciamo così, secondaria e in qualche modo accessoria

ognuno dei quali meriterebbe uno specifico dibattito parlamentare. Da una parte abbiamo la tragedia di un ragazzo, che forse è stato mandato con un po' di incoscienza a fare una tesi di dottorato e ad addentrarsi in materie di una certa complessità. Poi abbiamo una situazione, quella del Nord Africa, che andrebbe ripercorsa con maggiore profondità. Ma diciamo semplicemente una cosa, signor Presidente, tutti noi siamo stati testimoni degli entusiasmi provocati dalle cosiddette primavere arabe e poi siamo stati anche testimoni delle situazioni drammatiche che quella politica estera, che evidentemente era - diciamo così - un po' approssimativa, ha determinato. Abbiamo avuto anche contezza di quanto sia difficile esportare la democrazia e soprattutto il nostro modello di democrazia, sempre ammettendo che la democrazia sia il regime meno

che ha trovato una sua stabilità e un Governo che ha retto di fronte al rischio di un regime di tipo, diciamo così, religioso che avrebbe eliminato non soltanto la democrazia ma anche la laicità nello scontro politico. Poi, accanto a questo, abbiamo un terzo problema - sono tre problemi connessi - e cioè sappiamo perfettamente quanto profonda sia l'opera dei servizi deviati in Paesi già di per se instabili. Abbiamo, quindi, un oggettivo dubbio su come stanno operando e hanno operato quei servizi in Egitto per destabilizzare una delle poche teste di ponte stabili rimaste nell'area. Questo Parlamento deve decidere se questi tre problemi sono connessi tra loro e se si vuole mettere in connessione il dramma di Regeni con la situazione dell'Egitto, senza sapere quale sia stata l'attività dei servizi segreti, oppure se questi problemi mantengono una drammatica caso, un Parlamento serio non fa nemmeno lontanamente un emendamento, come quello che è stato presentato, per creare una connessione della quale non è certo in termini marginali, una scelta di politica estera che invece è fondamentale e che avrebbe avuto bisogno, in ogni caso, di un altro dibattito e di un'altra responsabilità da parte del Governo; non gli sguardi sulle carte e un po' di distrazione, scaricando sul povero relatore di turno una scelta di questa entità. *(Commenti del senatore Giovanardi)*. Questo è ciò che la serietà di un dibattito come questo avrebbe significato ed è per questo, signora Presidente, che il mio è un appello alla serietà. Il ritiro di questo emendamento e la sua sostituzione con un ordine del giorno, sul quale ci può essere la la completezza di un voto del Parlamento e magari anche l'unanimità, che rimetta le cose in ordine, senza operare forzature e indebiti collegamenti, sarebbe la cosa che più onorerebbe questo consesso.

Tuttavia, alla luce di come si è sviluppato il dibattito - e le chiedo scusa per essere stato aggiuntivo nel volermi sovrapporre prima in dichiarazione di voto a favore del subemendamento del senatore Tarquinio - prendo adesso la

La mia dichiarazione è contro questo emendamento. Come al senatore Quagliariello, anche a me farebbe piacere che il senatore Sangalli ritirasse

che attengono alla necessità di non allargare a una questione di pezzi di ricambio fondamentali scelte di politica internazionale; Quagliariello me lo consente, che ci sia qualcosa di più: c'è la dignità di una concezione di dottrina dello Stato. Gli Stati non sono associazioni a delinquere, fin dai tempi in cui Sant'Agostino si domandava cosa fossero, a proposito del pirata, che era tale perché lo faceva con un piccolo naviglio. Gli Stati non sono associazioni a delinquere e non hanno, tra i loro strumenti, l'allusione, il rancore e l'astio, trasferito senza assunzione di responsabilità

della presenza, se non del Presidente del Consiglio, del Ministro degli esteri e del Ministro della difesa) ha letto quel piccolo brano della relazione di accompagnamento al proprio testo, ha dimostrato con quanto cinismo e con quanta leggerezza è stato proposto questo emendamento. Non c'è cinismo e non c'è leggerezza, perché sono sicuro che nel collega Sangalli siano prevalse considerazioni relative alla vicenda Regeni (considerazioni che lo onorano), ma il parlamentarismo è soprattutto senso delle distinzioni. Proprio il rispetto del dolore della famiglia Regeni, proprio il rispetto della dignità che portò il Governo italiano a ritirare il proprio ambasciatore in una certa fase implicavano che le questioni non fossero sovrapposte e men che mai che un emendamento sui pezzi di ricambio potesse sovvertire ogni altra decisione parlamentare in materia di politica internazionale, di lotta al terrorismo, di nostra concezione dello Stato. Certo i diritti umani sono importanti, sono sacri,

che chiaramente non si riduce alla fornitura o meno di pezzi di ricambio e quant'altro. È una decisione seria, pesante sul piano della politica estera e militare.

Perché i Presidenti delle Commissioni non si alzano e spiegano all'Assemblea la vera

chiari cosa va a votare, perché lo fa e quali sono le conseguenze di un atto di questo genere, se sono conseguenze giustificate a fronte di una ragione di fondo che, se non è

fare tre brevi osservazioni. La prima osservazione, sulla quale nel dibattito sono emerse delle questioni e degli interrogativi, e sulla quale mi sento di intervenire

perché parte rilevante di ciò di cui parliamo è già a destinazione. Con buona pace di tutti, fermo restando il valore simbolico dell'emendamento presentato, voglio ricordare che parte di questi materiali sono sicuramente già stati consegnati. In questo senso, pur comprendendo l'atteggiamento del Governo che nel rivolgersi all'Assemblea si sottomette alla sua opinione, ritengo impropria la strategia del Governo perché l'Esecutivo, nel momento in cui il Parlamento applica una sanzione a un Paese con cui ha rilevanti rapporti,

dalle cose che scrivono i militanti del Partito Democratico al proprio segretario politico. Sul «Corriere della sera», rivolgendosi al caro segretario Matteo Renzi, Maryan Ismail, cittadina italiana di origine somala iscritta al Partito Democratico, fondatrice del circolo PD «Città mondo» di Milano e componente della segreteria metropolitana milanese, scrive: «Sono musulmana, laica e progressista. Mi considero parte di un Islam numericamente maggioritario, purtroppo finanziariamente inesistente e dunque totalmente inascoltato. Siamo chiamati a palesarci solo per fatti riconducibili al terrorismo islamico. Non siamo neanche iconograficamente pittoreschi: veli e barbe non sono nostri segni distintivi. non perdiamo occasione per urlare la nostra contrarietà alla visione ortodossa di un Islam dove politica e religione sono profondamente intrecciate, identificabile in quel wahabismo» - qui vorrei l'attenzione del collega Sangalli «della Fratellanza Islamica promosso da varie sigle nazionali e territoriali». Questa è la questione. Facendo tale scelta oggi esprimiamo l'attenzione del Parlamento e la preoccupazione perché il nostro Governo abbia una posizione virile nel rapporto con l'Egitto sul caso Regeni. Contemporaneamente ci immettiamo in un vero e proprio budello tortuoso i cui termini hanno portato in Egitto la messa al bando di un'organizzazione fatta di milioni di componenti. Il mio invito ai colleghi del Partito Democratico è a prestare estrema attenzione. Non facciamo gesti che possano far pensare che il nostro Paese si schiera

questi pezzi di ricambio sono ancora a casa nostra, dobbiamo mandarceli ovvero sono già andati nel 2015? Se qualcuno rispondesse magari uno voterebbe sapendo cosa vota.

che faceva rientrare un carabiniere dall'Uganda per difetto di copertura, perché c'erano le risorse per tenerlo in Uganda ma non per farlo rientrare. Allora, se i ricambi sono già in Egitto, vorrei che il presidente Tonini mi dicesse se è coperto l'onere di andare a riprenderceli, perché delle due l'una: o sono qui e dobbiamo mandarli oppure dobbiamo andare a riprenderceli. Vogliamo sapere, prima di votare, se sono lì o sono qui,

dopo le affermazioni dell'ex ministro della difesa Mauro - ripeto, non uno qualunque, ma l'ex Ministro della difesa - che dice che questi pezzi di ricambio sono già *in loco*, sono già stati consegnati...

ApI, E-E, MPL) e LN-Aut)* e approfitto della parola per informare i colleghi che questo materiale non è stato affatto consegnato, ma è imballato nel porto di Taranto.

ho un grandissimo rispetto per la discussione che si è svolta. È comprensibile che di fronte a un fatto così drammatico ci possano essere degli approcci diversi su come affrontare e gestire la questione.

registrare atteggiamenti e punti di vista diversi, ma il senso della nostra iniziativa è questo e su questa linea non deroghiamo perché la fermezza del nostro Paese è fondamentale. Noi, infatti, pretendiamo verità, senza voler in alcun modo

Io frequento Taranto con la stessa assiduità del senatore Latorre, eppure non sapevo assolutamente che i nostri pezzi fossero depositati in quel porto. E poi sostanzialmente, dopo gli interventi del senatore Caliendo e di un ex Ministro della difesa, dai quali apprendiamo la situazione nella quale ci troviamo, mi scusi, senatore Latorre, se non riusciamo ad avere verità, perché la verità da questo Governo non ci viene mai detta in quest'Aula, per cui il Parlamento non si può mai formare un'opinione e non riesce a capire cosa può decidere e cosa può votare. Questa è la situazione nella quale ci troviamo ogni volta a dover decidere. C'è soprattutto un dato fondamentale: siccome noi abbiamo atteso che la Commissione

Senatore Volpi, faccia concludere il senatore Di Maggio, che copre anche con la sua statura

forse potremmo contribuire ad un serio dibattito parlamentare.

con dei funambolismi dialettici, ha cercato di dirci che improvvisamente nel corso del pomeriggio, dopo ore ed ore di discussione, ha scoperto che nel porto di Taranto ci sono dei cassoni con dentro i pezzi di ricambio degli F-16. E ce lo dice il Presidente della Commissione difesa,

ha dato un segnale fortissimo, richiamando l'ambasciatore. E adesso ci viene raccontato che questo Parlamento, all'insaputa del Governo che si rimette all'Assemblea, ha bisogno di dare un'ulteriore segnale di nascosto. Questo emendamento io lo porterò all'ambasciatore egiziano e glielo farò leggere. Gli dirò che, grazie al nostro funambolismo legislativo,

il risultato di questo segnale e i suoi danni collaterali sono che non vogliamo più dare i pezzi di ricambio e che, per questo motivo, se li deve andare a cercare da qualche altra parte; sennò noi la lotta al terrorismo con l'alleato egiziano non la faremo mai. E questo non è un modo di fare politica estera. Sottosegretario Rossi, ci dica qual è la verità. Ci dica cosa va a raccontare all'ambasciatore egiziano, ci dica cosa diciamo all'Egitto su questo argomento. Non è possibile attivare un percorso di questo tipo.

Signora Presidente, abbiamo superato, credo con poca eleganza, lo scoglio di quell'emendamento. Le chiedo, attraverso la Presidenza, di sollecitare la presenza di un Ministro, ma non per un problema di maggioranza e di opposizione, perché la stessa cosa la facevo quando ero nella maggioranza. Non è possibile che ci siano delle non risposte e dei silenzi su temi che, presidente Casini, non riguardano sempre i pifferi e i sax. Quindi chiedo anche ai due Presidenti di Commissione, con la loro eleganza e moderazione, di sollecitare, magari attraverso canali informali, la presenza di un Ministro,

alla sorveglianza aerea degli spazi ad est dell'Alleanza, perché tale sorveglianza è chiaramente in funzione antirussa. Mettere batterie antimissilistiche e sorvegliare spazio aereo al confine con la Russia è sicuramente un segnale

Io vorrei però capire e chiarire un punto. Il testo del Governo annuncia la necessità di una spesa di 908.000 euro, di cui al comma 10, per coprire il periodo dal 10 maggio al 30 giugno. Le Commissioni riunite propongono che questo periodo sia allungato al 31 dicembre 2016. Non si aggiunge nulla dal punto di vista della spesa. Quindi, ciò significa: o che la prima spesa quantificata dal Governo era assolutamente esorbitante; o che si deve arrivare al 31 dicembre 2016 spendendo gli stessi denari, il che a me sembra un po' opinabile possa accadere. Quindi, ancora una volta e su un fatto puramente tecnico, non più politico, auspicherei che il Governo chiarisse come si può arrivare al 31 dicembre 2016 senza

un cacciamine - che non è stata impiegata in relazione a tutto quel tempo, entro il 30 giugno, e che ci è stata ancora ancora richiesta per la sorveglianza navale dell'aerea Sud dell'Alleanza. Le cinquantadue giornate in cui doveva essere impiegata nel primo semestre sono state spostate sul secondo semestre e questo non comporta evidentemente alcun ulteriore

senz'altro accetto la riformulazione del Governo, ma resto perplesso circa alcuni aspetti inseriti nell'ordine del giorno, con riferimento alla questione ONU, che appare alquanto pretestuosa, considerando il buon esito dell'istruttoria già avviata sul tema negli anni passati dai nostri Ministeri. Pertanto, in un secondo momento potrebbe essere utile tornare sull'argomento in una visione più sistemica. Oggi limitiamoci a rispettare gli impegni internazionali già ratificati dal nostro Parlamento.

con particolare riguardo a programmi aventi tra gli obiettivi la prevenzione, la protezione e il contrasto alla violenza sessuale sulle donne e le bambine, soprattutto quando usata con tattica di guerra, con tattica di guerra, la tutela e il rispetto dei loro diritti umani, nonché le misure a sostegno delle iniziative di pace promosse dalle donne in attuazione della risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite n. 1325 del 31 ottobre 2000

la portata rispetto alla parte interna e aumentandola rispetto alla parte relazionale con i Paesi e con le Nazioni Unite. Sull'emendamento 8.2 il parere è contrario.

guerra. Credo che quel tipo di violenza sia assolutamente da escludere e che non si debba nemmeno mettere come alibi l'eventuale idea che possa essere utilizzata come tattica di guerra. Io lascerei il testo

e che le donne bruciate sono oggetto di guerra e sono uno strumento. Quindi, ritengo che rimarcarlo non soltanto serva, ma chiarisca una verità storica.

corretto) è una proroga di sei mesi al Governo per l'esercizio della delega legislativa, come dice il testo stesso, per la riorganizzazione della Presidenza del Consiglio. Cosa c'entra questo con le missioni internazionali? Ecco perché mi dicevo: ci sarà una ragione per cui è stato tolto l'emendamento x1.2 (testo corretto). termine per l'esercizio della delega legislativa per il riordino della Presidenza del Consiglio. Che c'entra questo con tutto quello che dice il titolo pur aggiungendo al titolo: «proroga del termine per l'esercizio della delega legislativa»? Dove sta l'omogeneità alla quale ci ha richiamato più volte la Corte costituzionale che, in alcuni casi, ha fatto anche di più dichiarando incostituzionali norme in vigore da anni? in vigore da anni? Non era questo il Governo che cambia passo, che va veloce e di corsa, con il pugno, lo schiaffo e il salto mortale? No, quello era di cento anni prima, ma siamo lì! lì! Il Governo, appiccicandola ad una norma sulle missioni internazionali, chiede sei mesi di proroga per esercitare la delega. Si fa una delega in gran parte in bianco,

*(M5S)*. L'emendamento dimostra quanto abbiamo sostenuto nel corso del dibattito sulla legge delega sulla pubblica amministrazione e, cioè, la necessità di rivedere quella scellerata scelta fatta dal Governo di abolire il Corpo forestale dello Stato. L'emendamento dimostra

a uno spacchettamento, a uno smembramento di quelle funzioni. Forse, alla luce di questo emendamento, il Governo dovrebbe subito ritirare lo schema di decreto legislativo e impedire che sia approvato e si arrivi a un parere. L'Esecutivo si prenda sei mesi di tempo e rifletta su questa scelta. All'interno di quel decreto legislativo ci sono alcune misure interessanti, come la razionalizzazione di alcune risorse delle forze di polizia e di certi servizi,

Ma l'ampliamento dei termini per l'esercizio della delega non può avere alcun riflesso sui lavori di Commissione e sul termine previsto nella legge n. 240 del 2015, che è di sessanta giorni per l'espressione del parere da parte delle Commissioni competenti. E dico questo perché vorrei evitare che la discussione sull'emendamento in questione si ribaltasse nuovamente in Commissione e tornasse a essere sollevata una questione che invece non può essere sollevata. L'articolo 1 della legge Madia prevede che il Governo abbia dodici mesi, dall'entrata in vigore della legge - è stata il 28 agosto 2015 - per l'emanazione dei decreti legislativi. E, come noi sappiamo, molti e davvero complessi sono stati già emanati dal Governo, esaminati dalla Commissione o sono in corso di esame presso la Commissione. Il termine che viene riservato quindi con disciplina speciale rispetto ai termini previsti dall'articolo 139-*bis* del nostro Regolamento, ovvero venti giorni, più altri dieci concedibili dal Presidente del Senato in casi di particolare complessità - per l'esame dei decreti legislativi

il testo della legge Madia prevede che, nel caso in cui il parere non intervenga entro sessanta giorni, il Governo può emanare il decreto legislativo anche in assenza di osservazioni da parte delle Commissioni competenti, peraltro in una disciplina che, al contrario - e specialmente, appunto - riserva al parere delle Commissioni competenti un effetto particolarmente severo. Qualora cioè il Governo non volesse uniformarsi alle indicazioni provenienti dalle Commissioni competenti, dovrebbe tornare in Parlamento conferendo le proprie motivazioni circa questa inottemperanza.

Collega Crimi, sono sofisticata quanto lei. Siamo entrambi di origine siciliana e per questo mi permetto una battuta confidenziale: noi siciliani abbiamo la presunzione di avere un modo sofisticato di ragionare. So bene che lei si è rivolto al Governo chiedendo di utilizzare quel termine per ritirare il decreto-legge e ripresentarne un altro con diverse scelte e motivazioni. Ad ogni modo, mi è parso opportuno precisare

Chiediamo al Governo di essere parte più attiva, in quanto non possiamo più stare sempre a sentire ciò che dicono i nostri alleati. Non possiamo più dichiararci pronti ad andare via dall'Afghanistan e, dopo tre giorni, dire l'esatto contrario perché qualcuno ha cambiato idea.

anche se interessa poco a tutti. Non possiamo assistere all'ineffabile Alfano che ogni giorno ci racconta favolette sugli immigrati. Ormai ne arrivano a migliaia - troppi

Noi non reggiamo più. Dobbiamo sbattere i pugni in Europa rispetto a tutto questo. Non è possibile che l'Italia dia contributi enormi, spesso superiori a quelli di Germania e Francia, in termini di uomini, in tutto lo scacchiere mondiale

Siamo in grado di reggerli o fra poco scoppieranno tutte le nostre città? Questo è il dato reale. E, quando scoppierà il popolo italiano, che ha già tanti motivi per farlo, chi governerà questa situazione? Il Governo

Signor Presidente, il dibattito a momenti ha rasentato l'assurdo, perché ci siamo concentrati più sulla banda di Mogadiscio

approvino delle missioni le cui finalità poi vengono completamente stravolte. Il che sarebbe magari forse anche il male minore; ma, stravolgendo le finalità, si ottengono risultati esattamente opposti rispetto a quelli che si vorrebbero perseguire. Il traffico illegale

Ma anche quest'ultima missione, che serviva a contrastare l'illegalità, è finita per trasformarsi in una sostanziale operazione umanitaria volta a raccogliere profughi e naufraghi.

violato le intenzioni con cui è stata istituita la missione. Di più, se la missione fosse stata portata a termine, cioè con imbarcazioni in acque libiche che respingano immediatamente ogni clandestino, avremmo ottenuto che, nel giro probabilmente di una settimana, non ci sarebbero stati più alcun tipo di partenza e alcun tipo di sbarco sulle coste italiane, greche e maltesi, perché

l'obiettivo contrario rispetto a quello che si diceva di voler perseguire. Bene hanno fatto altri colleghi a stabilire che ci deve essere una fine a queste missioni, che costano tantissimo. Una portaerei, con tutte le dotazioni e il personale militare di Marina, ha dei costi altissimi. Se esse servono come deterrente per la sicurezza del Paese, il Paese se ne deve fare carico. Se devono servire, però, per altri scopi e per raccattare naufraghi, questo non può essere accettabile. Avevamo osservato quanto fosse grave armare Paesi che non danno garanzie di stabilità.

Abbiamo sentito leggere una relazione accompagnatoria secondo la quale sono già stati inviati, ma abbiamo anche sentito il Presidente della Commissione difesa affermare con totale sicurezza che sono ancora stivati nel porto di Taranto.

politiche estere dello scacchiere del Medio Oriente, potrebbe avere un'altissima dose di pericolosità. L'abbiamo fatto notare e speriamo che quanto abbiamo paventato non si realizzi. Continuiamo a notare un'incongruenza: sono state sostanzialmente bocciate tutte le proposte emendative in cui si diceva che non è il caso di rafforzare le difese antirusse della NATO,

sul posto, e non per contrastare il terrorismo, ma per tutelare gli interessi di una società italiana. A noi non dispiace che la società Trevi abbia

nei paraggi del cantiere operativo debbano essere caricati sul groppone dei contribuenti italiani. Non possiamo non notare che abbiamo votato un qualcosa che, a parere del Gruppo della Lega, che si è consultato in proposito, è anticostituzionale.

Può essere utile ma, secondo la dichiarazione della collega Finocchiaro, è pleonastico e non serve assolutamente a niente, perché le Commissioni riunite 1a e 4a hanno già iniziato l'esame del provvedimento di riordino. E, poiché scade a fine agosto, posso dire che abbiamo sessanta giorni di tempo nelle Commissioni e poi in Aula per convertire la delega del Governo. Pertanto, questa proroga potrebbe essere addirittura inutile, superflua e pleonastica.

le modalità di rapporto militare e non militare dei corpi volontari oltre che dei corpi militari della Croce Rossa, era stata allegata con la stessa facilità con cui era stato allegato questo emendamento,

diversi mesi fa abbiamo esaminato un provvedimento, meglio conosciuto come "legge quadro per le missioni militari all'estero", destinato a porre un freno alla decretazione di urgenza Grazie,

Sostanzialmente, rispetto agli anni passati non ci troviamo di fronte a delle novità: ancora centinaia sono i milioni destinati alle missioni armate e di molto inferiori sono le risorse per i progetti di cooperazione civile. E ancora una volta ci troviamo davanti alla decisione di aggregare in un unico provvedimento tutte le missioni militari all'estero, che invece hanno ciascuna una natura profondamente diversa. Vediamo le cifre. Per il 2016 sono 1,2 i miliardi di euro che il Governo destina alle missioni militari all'estero - la qual cosa costituisce una decisione in linea con quanto avvenuto lo scorso anno a fronte di solo 90 milioni (quindi meno 16 milioni rispetto allo scorso anno) per la cooperazione civile nelle stesse aree. ci troviamo di fronte a un decreto-legge, che quindi va approvato o respinto integralmente, seppure - ribadiamo - contenente missioni di natura e portata completamente differente. Questo ci fa riaffermare che, alla luce della legge quadro sulle missioni all'estero, che al momento si trova nuovamente all'esame dell'altro ramo del Parlamento, sarebbe stato più opportuno procedere con una suddivisione di queste missioni, tenendo conto della specificità territoriale e geopolitica, così da consentire al Parlamento di effettuare scelte più ponderate e rispondere già, ancorché attraverso lo strumento del decreto-legge, allo spirito della legge quadro che noi qui in Senato abbiamo approvato e che dovrebbe superare - speriamo a breve - il problema del raggruppamento forzato delle missioni. Tanto più che le missioni all'estero che questo decreto-legge va a prorogare sono rimaste prive di copertura giuridica e finanziaria, di fatto, per ormai i sei mesi trascorsi, dal momento che il precedente provvedimento di proroga è venuto a scadere il 31 dicembre 2015. Ma la cosa che mi preme mettere in evidenza è che nel testo oggi al nostro esame si esplicita solo la dotazione finanziaria dei diversi interventi, ma ben poco o nulla si specifica in merito all'ordine di ciascuna missione, per esempio - quali sono stati gli obiettivi raggiunti finora e quali quelli ancora da raggiungere; una programmazione, insomma, un obiettivo di politica militare ed internazionale. Alcuni contingenti dei nostri militari sono impegnati in talune missioni da più di un decennio. È, dunque, inevitabile domandarsi se questo provvedimento non riveli una carenza, che è quella del ragionamento sui risultati operati dalle nostre missioni e il punto sulla loro efficacia. II provvedimento in discussione, oltre a prorogare la missione in Afghanistan, che si sarebbe invece dovuta concludere nel 2014, continua a finanziare direttamente con 120 milioni di euro le forze di sicurezza di Kabul, sulle quali la comunità internazionale ha espresso forti riserve. Il tutto - ribadiamo - avviene senza un condizionamento degli importanti aiuti militari al rispetto dei diritti umani. Sui diritti umani, colleghi, noi non dobbiamo più transigere. Oltre a Libano, Kosovo, intervento antipirateria nell'Oceano Indiano, Albania, Palestina, Mali, area del Baltico per sorveglianza aerea, Bosnia e Cipro, il nostro Paese sarà anche protagonista della missione dell'Unione europea in Somalia, comandata da un generale italiano e a cui contribuiamo con un cospicuo contingente, per addestrare l'esercito locale. E tutto ciò avviene nonostante l'esercito somalo arruoli e utilizzi - secondo il Segretario Generale ONU - anche bambini soldato. Non è più concepibile. Occorre ritrovare la via del negoziato, perfino su diritti non negoziabili come quelli dei minori di non essere armati e coinvolti in conflitti di qualsivoglia natura. Notevoli risorse sono destinate a continuare l'impegno dei mezzi aerei in Iraq, mentre per ora non sono previsti fondi a favore della missione già annunciata di protezione del cantiere di una ditta italiana che dovrà ristrutturare la diga di Mosul. Questo costituisce uno dei punti che andava chiarito meglio. Il comma 9 dell'articolo 2 dice che è autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2016, la spesa di euro 236,402 milioni di euro con l'approvazione di un emendamento in Commissione è aumentata a oltre 253.875 milioni di euro - per la proroga della partecipazione di personale militare alle attività della coalizione internazionale di contrasto alla minaccia terroristica del Daesh. In questa cifra dovrebbero essere compresi, a decorrere dal 1° aprile 2016, sia un dispositivo di *personnel recovery* di 137 unità, sia un *team* di circa 100 militari incaricato delle attività propedeutiche alla *force protection* nell'area di Mosul, con particolare riferimento ai lavori di consolidamento della diga. Rispetto quindi alle due missioni in Afghanistan e Somalia potrebbe sorgere qualche interrogativo. Per la missione in Afghanistan, i 120 milioni di euro disposti al comma 3, articolo 9, per le forze di sicurezza di Kabul, vanno anche alla polizia nazionale afgana che, da più di cinque anni, viene messa nella lista nera dal Segretario Generale ONU nel suo rapporto su chi arruola e utilizza i bambini-soldato, crimine condannato dal diritto internazionale. Vorrei ricordare, inoltre, che il rapporto 2015-2016 di Amnesty International afferma che «sono state segnalate violazioni commesse dalla polizia locale afghana (ALP) fra cui intimidazioni, percosse, detenzioni illegali, uccisioni mirate, stupri di minori». Inoltre, il documento di Amnesty afferma che l'Afghanistan ha continuato ad applicare la pena di morte spesso al termine di processi iniqui. Per la missione in Somalia, i circa 25,582 milioni prevedono la proroga della partecipazione di personale militare alle missioni dell'Unione europea denominate EUTM Somalia. La missione ha l'obiettivo di contribuire allo sviluppo del settore della sicurezza con l'offerta di una formazione militare specifica, per 2.000 reclute somale. Secondo il rapporto del Segretario Generale ONU del 5 giugno 2015 «*Children and armed conflict*», le forze armate di Mogadiscio compaiono, come in passato, fra coloro che addestrano e utilizzano i minori in combattimento, in evidente spregio del diritto internazionale. Il Governo di Mogadiscio, anche secondo l'ultimo rapporto annuale di Amnesty International, è ritenuto responsabile di gravi violazioni dei più elementari diritti umani. Ricordiamo che l'Italia ha siglato nel 2013 un trattato di cooperazione militare con la Somalia finalizzato anche a rafforzare l'interscambio militare fra i due Paesi, nonostante la Somalia sia uno uno dei Paesi più poveri del mondo. In questo contesto, l'Italia dovrebbe subordinare ogni aiuto militare al rispetto dei diritti umani, in particolare ponendo fine, subito, al fenomeno aberrante dei bambini soldato. Anche per quanto riguarda la Libia i fondi sono cospicui, ma non è chiarita, e men che meno dettagliata, la ragione per la quale si è quadruplicato fino a 90 milioni lo stanziamento per la forza navale già impegnata. Questo Parlamento dovrebbe conoscere le finalità degli stanziamenti: si tratta non solo di danaro pubblico, ma anche di politica estera, il cui indirizzo non può e non deve essere misterioso. In sostanza, l'Italia è un Paese che a quelle latitudini sarà ricordato per la sua capacità di esportare modelli di democrazia, o come un mero erogatore di addestramento militare? Noi certamente ci auguriamo che questi profili di critica costruttiva vengano superati con la piena entrata in vigore della legge quadro sulle missioni e con i relativi decreti attuativi, perché diventi uno strumento valido per una corretta e completa discussione su ciascuna delle singole missioni. Ciò determinerebbe il necessario e serio impegno del Parlamento a dedicare la giusta attenzione alle missioni militari, che costituiscono un aspetto certamente fondamentale della nostra politica estera, che non è secondaria e senza conseguenze. Onorevoli colleghi, concludo auspicando che questo sia l'ultimo dibattito che il Senato svolge in assenza dell'operatività della legge quadro, dal momento che è necessario porre fine alla reiterata approvazione di decreti che dispongono solo finanziamenti decisi dal Governo in solitudine. Tuttavia, per consentire al nostro Paese di tener fede agli impegni internazionali assunti, dichiaro il voto favorevole del Gruppo Grandi autonomie e libertà, anche se, nel rispetto delle diverse sensibilità presenti all'interno del Gruppo, alcuni senatori esprimeranno un determinato e chiaro voto contrario.

Noi siamo convinti da sempre che le missioni dei nostri militari nelle aree critiche del mondo rafforzino l'Italia sullo scenario internazionale e siano anche un elemento di difesa dell'interesse nazionale. Dichiaro, quindi, subito il voto favorevole del nostro Gruppo Gli attentati di Parigi e Bruxelles hanno confermato la connessione stretta tra i conflitti in atto negli scenari di crisi e la sicurezza all'interno del Vecchio continente, dimostrando una volta di più la capacità operativa dei gruppi terroristici che sono in grado di operare sia nei teatri bellici tradizionali che nella guerra asimmetrica dentro le nostre città.

un particolare sforzo contro la minaccia del terrorismo. L'Italia sì è battuta perché l'area del Mediterraneo divenisse una priorità per l'Unione europea e per la NATO e, con Mare nostrum, ha salvato centinaia di migliaia di vite umane, ma ha raggiunto solo parzialmente il suo obiettivo. È vero che oggi c'è un impegno comune nel pattugliamento del Mediterraneo, con il proseguimento della missione EUNAVFOR Med, ma al doveroso salvataggio dei migranti che fuggono dalle guerre sono seguite né la redistribuzione dei profughi nei Paesi dell'Unione europea né una efficace lotta contro i trafficanti di uomini. insomma, sta facendo la sua parte di fronte a un fenomeno epocale come il flusso migratorio, ma l'Europa assolutamente no. Questo va detto ad alta voce, senza vantare successi che non ci sono mai stati da parte del Il Migration compact è una strategia di largo respiro, ma produrrà i suoi frutti solo nel lungo periodo. Quindi, ci vogliono interventi più efficaci a partire dalla revisione del Regolamento di Dublino. Non possiamo permetterci che 600.000 immigrati, attesi nel 2016 lungo la rotta mediterranea, restino tutti nel nostro Paese. Un'ultima considerazione: dal decreto-legge

Una situazione pericolosa, che potrebbe compromettere i nostri rapporti con Mosca proprio nel momento in cui il governo italiano si sta ponendo come ponte per la ripresa di una collaborazione più stretta tra Unione europea e Russia, soprattutto in funzione lo stesso ragionamento vale per il nostro contributo alla missione NATO "*Acrive Fence*" in Turchia. Dopo essersi schierata in chiave anti-russa, l'Italia sta valutando,

un bilancio rigoroso sulle dotazioni finanziarie, sul ripristino delle condizioni di pace, sull'eventuale miglioramento o - spesso - peggioramento delle condizioni economiche e sociali e degli *standard* democratici dei Paesi nei quali sono state costruite le principali missioni militari. Una per tutte continua per noi ad essere un terreno di forte polemica politica, quella in Afghanistan, rispetto alla quale, a fronte di un dal nostro punto di vista - fallimento militare, politico e sociale che si è perpetrato in quel Paese, non c'è mai stata in questo Parlamento una seria e adeguata riflessione

verso tutte le vittime civili, anche le ultime, quelle che, purtroppo, ieri sera, ancora una volta in una giornata drammatica, sono cadute

poi arrivano effettivamente nelle mani dei terroristi. Arriviamo al paradosso per cui noi combattiamo contro le armi che noi stessi abbiamo dato

riguarda i diritti umani, in particolare dei bambini soldato, crimine condannato dal diritto internazionale. Il decreto-legge in esame stanzia 120 milioni di euro per le forze di sicurezza di Kabul, Kabul, destinate alla polizia nazionale afgana, che - come tutti i rapporti ci dicono, anche quello del Segretario Generale dell'ONU sui Paesi che arruolano e utilizzano i bambini soldato

una questione così seria e drammatica che, non foss'altro che per questo terreno di serietà e di drammaticità, meriterebbe un approfondimento specifico di questo Parlamento e non di essere una

sull'emendamento, che peraltro parte da una nostra iniziativa politica e parlamentare, che propone di sopprimere le cessioni a titolo gratuito all'Egitto dei materiali di ricambio per i velivoli F-16. Pensiamo Pensiamo di poter dire che cogliamo in questo voto favorevole un segno positivo, che ci fa dire che non abbiamo voluto dimenticare

semplicemente elementi di solidarietà a parole e che invece bisognava mettere in campo elementi concreti e da questo punto di vista

attorno alla drammatica vicenda di Giulio Regeni, abbia ottenuto un elemento positivo. Naturalmente si tratta di un elemento positivo che però, inserito come è ovvio - in un contesto molto più ampio, che invece ci fa vedere ancora oggi una serie di perplessità e di contrarietà molto significative, comunque non ci mette in condizione di esprimere un voto diverso da quello contrario che, come abbiamo fatto in questi mesi, ribadiamo ancora una volta in questa sede

Vorrei ringraziare il Presidente della Commissione difesa e i relatori, che hanno svolto un lavoro impeccabile e le cui parole ci rappresentano in pieno,

internazionali di pace, delle Forze armate e di polizia, delle iniziative di cooperazione allo sviluppo. Sono venuto in queste ore dal Kurdistan, dove abbiamo non solo 500 militari, ma straordinarie opere della cooperazione allo sviluppo, di

non l'uso della forza fine a se stessa, ma l'uso della forza finalizzata alla pace, alla libertà di quei popoli e alla solidarietà alle persone che soffrono. Non desidero aggiungere altro, ma voglio dire che mi è sembrata impropria la polemica riguardo ad un atto simbolico che i relatori hanno proposto e che era sostanzialmente un segnale di disagio nei confronti dell'amico Egitto, perché l'amico Egitto è tale e i termini della questione non possono cambiare. Si è trattato, però, di un atto simbolico che dimostra come questo Parlamento non dimentichi e come la ricerca della verità per un connazionale barbaramente ucciso sia un atto di dignità e di decoro nazionale, soprattutto quando ci sono venute a più riprese spiegazioni inaccettabili, confuse e compromissorie di cui non abbiamo - noi sì - alcuna responsabilità e di cui hanno responsabilità le autorità egiziane. Ecco perché ritengo inutile questa polemica. Ritengo importante che si prefiguri un atto unitario del Parlamento e sono fiero che anche le forze di opposizione più responsabili vogliano concorrere con il loro voto ad un atto che deve unificare l'Italia e gli italiani. *(M5S)*. Signor Presidente, signori del Governo, onorevoli cittadini che ci ascoltate da fuori, fortunatamente ci siete voi perché qui ci saranno una decina di persone e non di più.

troviamo a discutere e, tra poco, anche a votare l'ennesima legge quadro che inorgoglisce il presidente Casini,

senza copertura finanziaria, giuridica e anche politica. Questa è l'ennesima dimostrazione che, dal punto di vista della programmazione, realmente il lavoro svolto dal Governo e da questa maggioranza è assolutamente pessimo.

i microfoni sono spenti, parlando con chiunque, concordiamo tutti quanti, però poi, alla fine, anche dentro questa Assemblea, vediamo una ipocrisia assolutamente inaccettabile. Mi rivolgo a tutti quei che hanno osteggiato, anche con veemenza, questo decreto-legge e che poi si troveranno a votarlo, con la scusa di appoggiare i militari. Ma qui non appoggiamo i militari e i lavoratori, appoggiamo le scelte scellerate di una politica estera e di difesa che non è quella italiana, è quella degli Stati Uniti

avete visto tutti quello che è accaduto ieri sera in Turchia - come può il Ministro prendersi la responsabilità di spostare 112 milioni su 245 (vale a dire quasi il 50 per cento) su altre missioni? È assolutamente inaccettabile! Ma andiamo avanti.

non rispettano minimamente le regole. Davanti a questo, l'Italia può prendersi la responsabilità di dire che a queste Nazioni non consegna armamenti perché quelle armi che oggi andrebbe a consegnare per uno scopo possono essere utilizzate dall'ISIS, anche contro l'Italia stessa? Possiamo prenderci questa responsabilità o no? Il Ministro dov'è? Perché non dà queste risposte?

- in cui si denunciano tutti i crimini che vengono perpetrati in Somalia, dove vengono utilizzati i bambini per la guerra.

non possiamo armare gli altri e avere la coscienza pulita nel dire che noi ripudiamo la guerra, mentre nel frattempo gli altri si scannano, si ammazzano. È assolutamente inaccettabile perché in questo

Bisogna iniziare da subito a parlare di un nuovo modello di difesa dell'Italia. Bisogna parlare di una difesa che sia sostenibile sostenibile per il DNA di questa Nazione, vale a dire l'accoglienza e non l'offesa. Va benissimo la difesa. Vogliamo una difesa che sia sostenibile, anche e soprattutto dal punto di vista finanziario. È inaccettabile che l'Italia porti porti avanti programmi come quello sugli F-35. Anche in questo caso, sfido chiunque a dirmi quanti F-35 sono stati prodotti. Siete andati a vedere con i vostri occhi quello che è stato prodotto nella base di Cameri?

euro che potevamo e dovevamo destinare ad altro. Cerchiamo di ridurre e razionalizzazione questa macchina, perché è assolutamente insostenibile. Andiamo a leggere il programma di questo Governo e di questa maggioranza, che si riempiono la bocca

che prima hanno votato contro alcuni emendamenti che avrebbero potuto ragionevolmente condividere e sostenere. Il presidente Casini ha detto di apprezzare la nostra responsabilità verso le Forze armate e i temi della sicurezza e delle missioni militari, che ci porta ancora oggi

del terrorismo, perché disarma chi in Egitto il terrorismo lo combatte, e alla vicenda di EUNAVFOR Med, che prima o poi si dovrà chiarire. Ma continuate così. Una delle ragioni di perdita di consenso dell'Europa, dei Governi europei e anche di Renzi è la politica suicida sul fronte dell'immigrazione.

che, in tante parti dell'Africa e dell'Asia, hanno offerto, anche adesso, un contributo al risanamento dei territori. Penso a quei nostri militari che in Afghanistan contribuiscono, con fatica e grave rischio, a consolidare delle istituzioni che - Dio lo voglia - prima o poi potranno essere autosufficienti, evitando il rischio che i talebani riconquistino quei territori. Ci sono tante altre missioni, piccole e grandi, che in tutta

di prorogare la missione in Afghanistan. Noi avevamo previsto questa necessità. Non siamo subalterni alle scelte degli Stati Uniti d'America e ci sarebbe molto da dire sul bilancio della presidenza Obama, dopo otto anni: un bilancio catastrofico. Basta vedere la mappa del mondo come era otto anni fa e come è adesso, l'avanzata del fondamentalismo islamico, la tragedia dello Stato islamico che occupa dei territori, gli errori di valutazione sulle primavere arabe e quant'altro. Noi avevamo previsto che si sarebbe dovuta prorogare la missione in Afghanistan, perché un ritiro intempestivo avrebbe facilitato una riconquista da parte di talebani e fondamentalisti. Oggi, rispetto agli anni di Al Qaeda, il fondamentalismo ha fatto dei passi in avanti perché ha conquistato dei pezzi di territorio. Al Qaeda, pericolosissima organizzazione criminale e protagonista di efferati attacchi anche al mondo occidentale, oltre che nelle aree arabe e asiatiche, ha visto il suo superamento, perché lo Stato islamico, rispetto ad Al Qaeda, ha pezzi di territorio, banche e pozzi petroliferi. l'esame di questo provvedimento, qualche ordine del giorno e qualche osservazione che abbiamo avanzato noi e i colleghi della Lega hanno riguardato anche gli errori che si fanno nei confronti della Russia, con manovre della NATO come se fossimo di fronte alla Russia sovietica degli anni Settanta. L'epoca dei blocchi e della contrapposizione giustificava un atteggiamento guardingo e difensivo.

nell'impotenza. Noi diamo sostegno e solidarietà ai nostri militari, che partecipano a queste missioni, e riteniamo che l'Italia abbia anche ulteriori doveri da affrontare. Vedremo come evolveranno

stanno difendendo la legalità e la democrazia. A questi diamo un voto favorevole, ma non ad un Governo, presidente Casini, che anche oggi si è distinto in maniera assurda. Voglio ribadire le ragioni che ci lasciano amarezza nel votare a favore, guardando a quell'Italia di fierezza e di legalità, che dà un contributo anche alle popolazioni. Si è discusso, in Commissione e in Aula, se queste missioni diano anche un soccorso alle popolazioni. Ma certo che lo danno; ovunque pasti e assistenza medica. Avremmo potuto - lo dico alla Presidenza - forse anche varare quelle norme sul corpo della Croce Rossa che sono comunque necessarie, Croce rossa il cui smantellamento a tappe non abbiamo

Regeni in Egitto non hanno fornito i necessari elementi di conoscenza e di verità sulla loro corresponsabilità. Cosa era stato mandato a fare? A quali rischi è stato esposto quel ragazzo? Questa mattina ho letto anche i nomi. Ho apprezzato le parole del senatore Giuseppe Esposito, tuttavia il suo Gruppo non l'ha seguito. Non ho visto il senatore avreste potuto meditare su quello che lui, da vice presidente del COPASIR, ha detto.

senatore Latorre, protagonista del processo di modernizzazione della sinistra italiana, oggi ci ha dimostrato che è stato comunista anche lui, perché, con qualche reminiscenza,

XVII).* Lo so che la sua era una battuta, perché non fa queste perizie. Si possono dimostrare in mille modi le posizioni italiane sul caso Regeni e chiedere la verità, ma non, all'indomani dell'attentato di Istanbul, disarmare l'Egitto che combatte contro il terrorismo. E noi, pur criticando la reticenza sulla vicenda Regeni ed esigendo la verità, La fase tre non scatta, la fase due prosegue, continuate così. Avete la direzione

un ritorno costante ed esponga anche al rischio talvolta, per via dei ritardi che anche oggettivamente si possono determinare, di avere momenti di scopertura

questo rito che - ahimè - da molto tempo va avanti, con decreti‑legge che di volta in volta non consentono di fare una discussione forte e programmatica rispetto agli impegni internazionali del Paese per poi delegare il Governo alla gestione pratica di questi passaggi.

in uno scenario molto problematico, in cui l'offensiva terroristica continua ad essere molto pericolosa e molto preoccupante. Penso a quello che è accaduto in queste ore in Turchia e approfitto di questa occasione, dopo che questa mattina abbiamo dedicato un minuto di raccoglimento, per ribadire la solidarietà e la vicinanza nostra e credo di tutto il Parlamento alla Turchia, a quel popolo e anche a quel Governo.

tanto più in un momento in cui anche il progetto europeo è esposto a quei rischi e a quelle difficoltà segnalate anche dall'esito del *referendum* britannico. Non dimentichiamo che la Gran Bretagna è un *partner* fondamentale delle nostre politiche di sicurezza e di difesa e che dunque questa decisione inglese ci impone di accelerare un processo di costruzione del sistema europeo di difesa.

è stato prorogato di un anno e oggi finalmente, anche alla luce della risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, è un programma che consente di addestrare, da un lato, la guardia costiera e la componente marittima dell'esercito libico sostenuto dal nuovo Governo e, dall'altro, di controllare le acque e tutti i traffici che attraverso quelle acque

missione è in contraddizione con questa esigenza e con questa priorità. Vorrei anche dire, tanto più alla luce di quella indagine conoscitiva, caro collega Santangelo, che anche in virtù della vostra iniziativa abbiamo portato avanti e che

di un assetto del sistema di difesa e di un ruolo del nostro Paese che si colloca in una dimensione internazionale e che assume il tema della missioni come prioritario obiettivo di quel lavoro di *peace keeping* e addirittura di *state building* che sta consentendo di costruire un modello italiano vero e proprio, al quale guardano anche gli altri Paesi. Certo, questa politica e questa idea dell'assetto del sistema di sicurezza e di difesa in alcun modo possono venir meno al principio principio che pace e sicurezza sono due facce della stessa medaglia, e che non c'è nessuna politica per la pace che prescinda anche dalla capacità di garantire la sicurezza delle nostre società. Questi sono due ingredienti fondamentali, che devono andare di pari passo. Un grande Paese come il nostro non può in alcun modo andare oltre quel confine che separa la politica dalla testimonianza, perché un sistema di difesa e una politica della sicurezza non possono esplicarsi soltanto in una testimonianza, ma devono esplicarsi nel saper combinare

di entrare nel merito di alcune questioni, da ultimo, sull'emendamento sul caso Regeni. Come è stato opportunamente precisato anche dal collega Casini, presidente della Commissione esteri, ha, il significato di voler ribadire una volontà e un impegno, che non compromettono le relazioni con quel Paese, ma che pretendono verità. E vorrei dire al collega Romani, che vuole portare il testo di quell'emendamento all'ambasciatore egiziano, che, quando lo farà, gli dica che questo Parlamento vuole la verità sul caso Regeni. Glielo dica e glielo ricordi. Per concludere,

e per attuare una politica internazionale adeguata alle nuove difficoltà e alla natura nuova delle crisi e dei conflitti. Questo vale soprattutto in tempi difficili come quelli che stiamo vivendo. Le tensioni le emergenze sociali ed economiche rendono più difficile spiegare perché impegniamo risorse in missioni così lontane. In realtà, esse così lontane non sono e lì si gioca la partita decisiva anche per la nostra sicurezza, per la pace e per il futuro del nostro Paese. Con questo spirito e con queste determinazioni noi daremo il nostro voto favorevole a questo provvedimento.

il ruolo dei libici, del Fronte di liberazione della Palestina e dell'autonomia, quando organizzò e preannunciò una rappresaglia contro gli innocenti, proprio nel giugno del 1980. Perché queste cose non si devono sapere? Perché non si devono approfondire? Vedete, perché mi astengo? Perché, se fosse vero quello che tanti di voi dicono, che la Francia e gli Stati Uniti sono bugiardi e assassini, come viene detto pubblicamente e viene cantato a Bologna negli spettacoli, perché allora il Governo italiano, in questo Parlamento che applica le sanzioni all'Egitto, tace totalmente con gli Stati Uniti e con la Francia? Perché nessuno solleva il problema rispetto a Governi che sono accusati di aver assassinato 81 nostri innocenti concittadini? Perché non si prendono iniziative? Ve lo dico io: perché noi siamo forti con i deboli e deboli con i forti e arriviamo a dei risultati che sono di viltà - lo devo dire al Governo - anche grotteschi. Apprezzo che il Governo abbia detto al Parlamento «mi rimetto al Parlamento», ma mi sembra vile e grottesco l'atteggiamento di un Parlamento che mette a rischio la lotta al terrorismo internazionale dando uno schiaffo in faccia ad un nostro alleato e nel contempo tace rispetto a una cosa che secondo me è lunare, rispetto alla bomba che sarebbe stata messa e che sarebbe stata coperta. Nessuno vuole andare a vedere le carte segrete che raccontano un'altra storia, ma nel contempo non dice una parola nei confronti di Governi che ogni giorno vengono accusati di essere complici di quell'infamia. Ditemi se questo è il comportamento di un Parlamento! nel silenzio assoluto di tutti. *(Commenti dal Gruppo PD)*. Ad oggi nessuno, tra tutti coloro che sono intervenuti, ha chiesto di togliere il segretissimo o ha chiesto di fare luce e verità. Chiediamo all'Egitto di fare luce e verità su quell'accadimento, ma non chiediamo al nostro Governo di togliere il segreto su vicende che riguardano 81 cittadini

Prima di procedere alla votazione finale, avverto che è stata presentata dal relatore Vattuone, ed è in distribuzione, la proposta di coordinamento C1. Poiché tale proposta interviene sulla copertura finanziaria, chiedo al presidente della Commissione

Signor Presidente, con questo intervento di fine seduta inizio oggi al Senato una staffetta con cui, assieme a tante altre senatrici, ricorderemo ogni donna che verrà uccisa per mano di un uomo a cui è o è stata legata da relazione amorosa. Lo faremo fino a che sarà necessario ricordare al Parlamento e al nostro Paese l'urgenza di arginare la violenza nei confronti delle donne. Lunedì notte, a Modena, una donna, Bernadette Fella, è stata uccisa dall'ex convivente. Martedì notte è stata la volta di Manuela Precerutti, uccisa a Dorno, a Pavia, dal compagno davanti alla figlia. Secondo la stampa si è trattato di una "tragedia della follia" a fronte di un "amore tormentato". L'ISTAT ci informa che in Italia ogni 2,2 giorni viene uccisa una donna e che il 46,3 per cento delle donne muore per mano del *partner*. La gravità delle violenze sessuali e fisiche è aumentata e sono in crescita anche i casi di violenza assistita. Sui media la violenza sulle donne è quasi sempre descritta come frutto di motivi passionali, lo stereotipo dell'amore tradito che giustificava il delitto d'onore si trasforma in quello della gelosia, del tradimento, dell'abbandono che l'uomo non è stato in grado di accettare. L'uomo è quindi da compassionare, il suo è stato un gesto estremo (un *raptus*). Una spiegazione, insomma, che dando un'attenuante al colpevole, addossa alla donna una parte di responsabilità in quanto colpevole di avere suscitato la gelosia. Si tratta di una rappresentazione falsata della realtà. Il femminicidio è quasi sempre l'estremo risultato di una serie di comportamenti violenti di lunga data. Con la legge n. 119 del 2013 di contrasto alla violenza di genere che questo Parlamento ha approvato in attuazione della Convenzione di Istanbul, il nostro Paese ha riconosciuto la violenza sulle donne come violazione dei diritti umani e discriminazione di genere, ha riconosciuto che la violenza sulle donne è un fenomeno sociale che ha le proprie radici nella relazione di potere, asimmetrica tra uomini e donne. Per questo la si può prevenire, intervenendo sui fattori che la determinano. Per questo è stato proposto e approvato un piano contro la violenza sulle donne. Nel frattempo sono stati rafforzati strumenti di protezione per garantire maggiore sicurezza alle donne minacciate. Bisogna, però, monitorare affinché queste misure funzionino e che il piano sia attuato. Bernadette Fella aveva denunciato le violenze subite nel 2012; il processo verrà celebrato nel settembre 2016; l'altra notte è stata ammazzata. Cosa non ha funzionato nella rete di protezione? Un appello alla Ministro per le pari opportunità e al Governo tutto: si monitorino l'applicazione, i pregi e i limiti della legge n. 119 del 2013 e soprattutto si dia piena e accurata attuazione al piano contro la violenza. Un appello ai *media*: si smetta di giustificare gli assassini e di colpevolizzare le donne. Un appello al Paese, uomini e donne: sono 160 le donne uccise ogni anno. Non possiamo più accettare questa mattanza.

nelle città da Francavilla al Mare fino a San Salvo, in tutta la costa chietina, le vongole non crescono più di 11

una delle più belle spiagge d'Italia, inquinato per colpa del fiume Pescara. Di fronte a ciò nessuno fa niente, le depurazioni sono a zero. Penso che il Governo debba dare una risposta. I Ministri dell'ambiente e dell'agricoltura

ho chiesto da molti mesi che il Governo riveli un fatto che è di interesse certamente pubblico: chi ha firmato i provvedimenti che hanno autorizzato la società A4, che gestisce l'autostrada Brescia-Padova, a a prorogare la presentazione di determinati documenti funzionali alla continuazione della concessione, che frutta oltre 300 milioni all'anno di incassi, circa metà dei quali sono di profitto.

dato. Sarebbe interessante sapere chi, arbitrariamente, modificando un atto che è stato approvato anche dal Parlamento, ossia la convenzione del 2007 tra l'ANAS e la società A4, ha concesso a questa società privata di farsi un guadagno di un miliardo. il Governo, dopo lunghissime sollecitazioni, è finalmente venuto a rispondere a questa interrogazione e non ha detto né il nome della persona che ha firmato, né quanti sono gli atti, né quando sono stati firmati; firmati; non si sa neppure se l'atto è stato firmato sotto la responsabilità del Governo Monti o del Governo Letta, essendovi stata la prima firma nel 2013;

agli atti previsto dalla legge n. 241 del 1990 e il Ministero non ha risposto. Ho fatto ricorso alla commissione per l'accesso, la quale ha detto che il parlamentare non ha diritto all'accesso perché ha già le interrogazioni, ma il Governo non risponde. Intanto chiederò al Governo che utilizzi la delega proprio per modificare la legge sull'accesso, chiarendo questo aspetto. Nel frattempo io interesserò della questione l'Autorità nazionale anticorruzione, perché se il Governo non vuole rivelare l'identità di chi ha redatto una firma che costa un miliardo al contribuente italiano, evidentemente è perché c'è qualche conflitto d'interessi o peggio ancora. Pertanto a questo punto è una questione che con mio rincrescimento devo affidare ad autorità di carattere giudiziario o paragiudiziario, visto che le prerogative parlamentari vengono calpestate e irrise dal Governo.

La notizia non è stata riportata solo da quel giornale, ma da tante testate nazionali e anche da RAI2 all'ora di pranzo. Ebbene, io ho contattato direttamente l'ospedale Gaslini di Genova e questa notizia che riferisce di una bambina che sarebbe finita in rianimazione a causa dell'alimentazione vegana della mamma (quindi anche della bambina che ha un anno) in realtà non è veritiera, perché, proprio come riferitomi circa un'ora fa dal direttore sanitario dell'ospedale Gaslini di Genova, risulta che la bambina, durante l'alimentazione dei primi mesi di vita dopo lo svezzamento, avrebbe assunto anche parmigiano. Ovviamente, come potete immaginare,

quindi probabilmente la mamma non seguiva una dieta vegana con tutti gli accorgimenti del caso. Non solo, ma questa notizia, oltre a essere falsa, è l'ennesima strumentalizzazione. Infatti, basterebbe pensare al 15 ottobre dell'anno scorso, quando su «Il Gazzettino» di Treviso era apparsa la notizia di un bambino in ospedale perché vegano. Ebbene, anche in quel caso contattai il direttore sanitario dell'ospedale di Treviso e proprio in quel frangente mi fu riferita la stessa circostanza, cioè che il bambino aveva